da parte di 769 detenuti «fine pena mai» e di 13.000 sottoscrittori del loro appello.

quanto accaduto qui giovedì scorso su questioni di procedura, non di sostanza, perché non mi permetterei di utilizzare il richiamo all'ordine dei lavori per introdurre un dibattito di merito.

e di inammissibilità. Probabilmente questa dichiarazione già avrebbe dovuto esser fatta dal Presidente della 1a Commissione permanente; tuttavia, il fatto che il presidente Bianco non abbia esercitato questa facoltà non significa che non possa essere esercitata dall'Aula. Tra l'altro, Presidente, ricordo che in materia di decretazione d'urgenza vi è un parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984 cui si ribadisce, in particolare per i decreti-legge, che occorre che gli emendamenti siano collegati ai temi, agli argomenti e alle materie trattate dal decreto-legge, cosa che non si è invece verificata famoso emendamento sull'omofobia, né per altri emendamenti che trattavano argomenti assolutamente diversi. Le ricordo, Presidente, che nella prassi parlamentare quantomeno ci si preoccupava di individuare nel decreto-legge una norma - che veniva definita "rampino" - per poter ricollegare materie che altrimenti sarebbero state estranee e, quindi, dichiarate inammissibili. Credo che questa questa abdicazione a una sua facoltà, a una sua potestà e a un suo obbligo alla fine si sia ritorta, Presidente, contro la funzionalità e contro la stessa funzione politica che lei esercita: nel decreto‑legge è entrato un argomento così estraneo a quella materia che ha dato luogo - direi giustamente - ad una rivolta anche di coscienza da parte dei senatori della maggioranza nella quale lei si riconosce. Né, Presidente, vale a superare questa obiezione il fatto che, trattandosi di voto di fiducia, ci si debba coprire le orecchie, gli occhi e la bocca come le famose scimmiette perché lei ha sempre intatte le

questo principio a tutti i maxiemendamenti del Governo creeremmo delle leggi *monstrum* dove si potrebbe inserire qualsiasi tema e qualsiasi materia mai discussa, mai affrontata mai delibata dalla Commissione e dall'Aula, ma pur tuttavia oggetto di un voto del Parlamento con valore e forza di legge. Ricordo, Presidente, che un anno fa si sollevò questo problema; lei si impegnò ad affrontarlo

quando si è verificato un episodio spiacevole che ella, probabilmente, non avrà seguito, ma che ormai saprà perché è su tutti i giornali: l'aggressione avvenuta nei confronti della sottosegretaria Lucidi. Signor Presidente, è da tempo che in questo luogo - che merita che merita davvero rispetto perché è l'Aula del Senato - si verificano episodi di aggressione verbale.

se non fossero intervenuti i commessi ‑ che ovviamente ringraziamo ‑ non so se la sottosegretaria Lucidi non avrebbe preso

della Sottosegretario, in quanto membro del Governo e del Parlamento, ma in quanto donna. Già altre volte si sono verificati episodi di forte aggressività verbale, nei confronti, ad esempio, della

perché il Governo non è stato capace di dare una risposta alle questioni poste dagli autotrasportatori. Il ministro Bianchi è famoso perché il 25 maggio 2006 disse che ascoltando Fidel Castro provava una fortissima emozione. Spero che si sia rimesso da quell'emozione e la invito a sollecitare la sua presenza urgentissima in Parlamento perché - ripeto - il Paese si sta fermando. È vero che noi abbiamo le auto blu e quindi non dobbiamo preoccuparci di andare a fare benzina; è vero che abbiamo il ristorante del Senato e quindi non dobbiamo fare la spesa, ma, in questo momento, nel Paese sta mancando la benzina,

cosiddetto decreto espulsioni, vorrei ricordare un altro aspetto. Il presidente Pera era intervenuto durante la seduta facendo notare che il riferimento all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam

viene cancellata una serie di reati, come l'incitazione alla discriminazione per motivi razziali e per altre ragioni, la discriminazione per motivi razziali e altri motivi e addirittura gli atti di violenza per motivi razziali, religiosi, nazionali o etnici.

perché ritengo occorra ascoltare anche la controparte: per troppi mesi, questo Governo ha rifiutato l'incontro con la controparte ed oggi ci ritroviamo con l'Italia paralizzata.

su un altro *dossier* importante che si sta discutendo in queste ore. Ciò che lascia perplessi noi parlamentari è che questo*dossier* viene discusso all'esterno delle sedi competenti, mi riferisco alla vicenda Alitalia che è particolarmente delicata. Ora, noi avevamo già sollevato in quest'Aula la

Onorevoli colleghi, sono certo di interpretare il sentimento di tutta l'Assemblea dedicando, all'inizio dei nostri lavori, un momento di riflessione e di raccoglimento per ricordare i quattro operai periti nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino la scorsa settimana e con essi le centinaia e centinaia di donne e uomini che, anche quest'anno, hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Giovedì verranno celebrati i funerali ed il Senato sarà presente con una sua delegazione, come l'Aula ha chiesto. Ieri, giornata di lutto cittadino a Torino, ho inviato al sindaco Chiamparino un telegramma per manifestare l'autentica vicinanza del Senato al dolore della città e, in particolare, dei familiari delle vittime. Dinanzi al rinnovarsi quotidiano di queste tragedie tutto il Paese si sente sprofondato in un sentimento di dolore, di angoscia e di rabbia. Altre volte, purtroppo, nei mesi recenti ho dovuto pronunciare in quest'Aula parole di ricordo di vittime del lavoro e di vicinanza ai loro familiari. Strage, piaga sociale, emergenza, queste sono le parole che usiamo per indicare lo stillicidio quotidiano di vittime. Credo però che un incidente così grave, in una realtà sociale come Torino, dove l'industria ha una sua radice culturale antica e dove tutto il contesto non può dirsi proprio impreparato, è una cosa ancora più seria ed inquietante. Il prossimo 1° gennaio celebreremo i primi 60 anni di vita della Costituzione, una Costituzione che ha sancito che la nostra Repubblica democratica è fondata sul lavoro. Ecco, io credo sia giunto il momento di compiere uno sforzo in più se, dopo tanti anni di impegno dello Stato, la piaga dei morti sul lavoro è ancora così grave. Dobbiamo assumere decisioni più incisive e profonde: è un dovere. La insufficiente sicurezza del lavoro si accompagna infatti ad una condizione di insufficiente qualità del lavoro, di non adeguata stabilità, di vera e propria precarietà, di formazione ancora troppo debole e di una cultura positiva del lavoro che deve riproporsi ed interpretare quei valori di responsabilità e di inclusione sociale che il lavoro storicamente contiene. Occorre che tutto il Paese reagisca, ognuno deve fare la sua parte. Il Parlamento, nei mesi scorsi, ha approvato il Testo unico sulla sicurezza; abbiamo istituito una speciale Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro; il Senato si è impegnato con largo consenso nel fare la sua parte. Servono altre leggi? Le Camere non si tireranno indietro, ne sono certo; è stato detto, però, che occorre applicare innanzitutto quelle che già esistono, allora si faccia con fermezza, senza sottovalutare, controlli e procedure essenziali per garantire le soglie di sicurezza. Credo che sia necessaria una forte cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, un'azione energica affinché nei luoghi di lavoro siano non solo salvaguardati, ma modernamente promossi i diritti dei lavoratori. La sicurezza è prevista nelle leggi e dobbiamo forse meglio saper individuare le responsabilità di chi concretamente non le applica. Ma la sicurezza è anche il risultato di una cultura complessiva, in una società che deve essere competitiva - le leggi di mercato ce lo impongono - ma non deve divenire violenta nei fatti. Una grande opera di sensibilizzazione, di informazione e di formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'opinione pubblica del Paese possono, tutte assieme, fornire una risposta concreta per sconfiggere questo flagello. Noi oggi ricordiamo i morti sul lavoro, ma non dobbiamo e non vogliamo dimenticarli domani, questo è il problema, per rispetto ad essi, ai loro famigliari e perché sappiamo che un'attenzione non episodica e frammentata potrà contrastare irregolarità, negligenze, illegalità. Penso anche che sarebbe necessario porre attenzione alle famiglie delle vittime, che non possono essere lasciate sole dallo Stato e dalla società.

Presidente, onorevoli senatrici e senatori, con riferimento a quanto accaduto presso l'acciaieria ThyssenKrupp, desidero esprimere tutto il mio cordoglio, anche a nome del Governo, alle famiglie degli operai coinvolti nell'incidente avvenuto presso le acciaierie torinese. Siamo di fronte ad una vera e propria strage nel lavoro, una strage di persone innocenti. Tutto questo ci lascia Tutto questo ci lascia sgomenti, anche perché l'incidente è avvenuto in una grande impresa, una multinazionale, un'impresa sindacalizzata, un'impresa con i delegati rappresentanti della sicurezza, non in un'impresa invisibile del sottoscala o del lavoro nero. Premesso il doveroso riserbo dovuto ogni qual volta siano in corso gli accertamenti penali, sul tremendo episodio posso dire quanto segue.

ha proceduto a nominare due consulenti tecnici con il compito di ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente. Allo stato attuale, le principali ipotesi ricostruttive dell'evento, descritto «come un'onda di fuoco che si è rovesciata sui lavoratori», riconducono la causa alla rottura di un flessibile che ha causato la fuoriuscita di olio sotto pressione o ad un piccolo focolaio alimentatosi con l'acqua. Attualmente sono in corso accertamenti su tutta l'impiantistica presente nello stabilimento, salvo la linea interessata dall'incendio che è posta sotto sequestro. In attesa dell'esito delle indagini in corso da parte della magistratura e della competente ASL si è stabilito il fermo produttivo dello stabilimento. Ogni possibile ripresa delle attività produttive è subordinata, comunque, agli esiti del negoziato sindacale delle parti. Credo che questo episodio richiami a tutti una discussione sul lavoro, sulla perdita della sua centralità, sulla sua invisibilità, sulla solitudine dei lavoratori, soprattutto quando parliamo di lavoro operaio e soprattutto sul fatto che quando parliamo di sviluppo dobbiamo insistere sulla qualità dello sviluppo che vuole anche dire qualità non solo della risorsa umana, ma anche qualità della sicurezza sul lavoro. che la nostra storia è stata costellata da incidenti mortali, da stragi sul lavoro. Se vogliamo andare ad un ricordo statistico, nel lontano 1963 ci furono in Italia ben 4.644 morti sul lavoro; se torniamo ai tempi più recenti, nel 2002, 1.481 furono le morti sul lavoro e l'anno scorso ben 1.302. Per noi, al di là degli andamenti delle statistiche, anche solo un morto sul lavoro è questione di costernazione, di disagio e di dolore da parte delle comunità interessate. Quello che vorrei riportare in questa discussione come il Governo ha inteso muoversi con interventi di carattere organico che hanno riportato al centro dell'azione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche sovvertendo quel senso di rassegnazione, talvolta di accettazione fatalistica che si è spesso registrato in occasione delle cosiddette morti bianche. La sensibilità e la profonda attenzione del Presidente della Repubblica Repubblica sul tema costituiscono un conforto ed un impulso nella direzione su cui il Governo si è mosso. Al fine di fornire un quadro molto sintetico sugli interventi normativi, vorrei ricordare, in primo luogo, la legge n. 248 del 2006 che, all'articolo 36-*bis*, riporta: «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro». Già nel 2006 abbiamo previsto: la possibilità di sospendere i cantieri dell'edilizia in caso di presenza di almeno il 20 per cento di lavoratori al nero; l'obbligo dei datori di lavoro di munire tutti i lavoratori edili di una tessera di riconoscimento; l'obbligo della comunicazione antecedente a quello della instaurazione del rapporto di lavoro per i datori di lavoro dell'edilizia; l'inasprimento delle sanzioni per la omessa iscrizione nei libri obbligatori dei lavoratori; la reintroduzione delle indennità di trasferta in favore del personale ispettivo, abrogata con la finanziaria del 2006. L'efficacia di questo provvedimento si può riscontrare nei seguenti dati per quanto riguarda il settore dell'edilizia che, come tutti sanno, è il settore unico di competenza per la sicurezza sul lavoro del mio Ministero. In dal mese di agosto 2006 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 ottobre 2007, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Il provvedimento di sospensione e di chiusura dell'attività ha riguardato nei quattordici mesi 2.829 imprese. È interessante sottolineare che nelle aziende destinatarie del provvedimento di sospensione erano impiegati il 61 per cento dei lavoratori in nero rispetto al totale dei lavoratori regolarmente occupati.

e un saldo contributivo, per quanto riguarda i contributi pensionistici, pari ad oltre 57 milioni di euro. Sempre in edilizia, in questi quattordici mesi, secondo la segnalazione dell'INAIL, ci sono state 189.000 assunzioni di nuovi soggetti non conosciuti dall'Istituto, di cui 84.000 italiani e ben 104.000 stranieri;

all'immissione di 300 unità di personale ispettivo risultato idoneo al concorso pubblico, per un totale, con queste unità, di 1.411 nuovi ispettori del lavoro assunti nei Inoltre, abbiamo previsto l'estensione a tutti i settori produttivi del documento unico di regolarità contributiva anche come accesso ai finanziamenti a favore dell'impresa. Abbiamo introdotto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative già previste per la violazione di norme in materia di lavoro e più gravose sanzioni in caso di omessa vidimazione ed istituzione di libri obbligatori. Vi sono poi state misure volte a promuovere l'emersione del lavoro nero e anche misure di stabilizzazione per favorire la trasformazione da lavoratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto in lavoro a tipo subordinato. Dai primi dati in nostro possesso risultano stabilizzati in questo periodo circa 22.000 lavoratori. Come previsto dai commi 1175 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa le modalità di rilascio dei contenuti del documento unico di regolarità contributiva. Inoltre, il 2 luglio 2007 si è provveduto a determinare l'importo destinato al fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Tutte queste misure si sono già evidenziate prima ancora di emanare, il 3 agosto 2007, la legge n. 123, che reca misure in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda queste ultime disposizioni, vorrei rapidamente ricordare che la legge si compone di 12 articoli, 11 dei quali già operativi dal mese di agosto di questo anno. Il primo articolo è di delega. La delega prevede: l'estensione del campo di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai lavori autonomi e parasubordinati; la semplificazione degli adempimenti in carico alle imprese; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio; la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza mediante la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi ispettivi; la formazione, intesa come strumento di prevenzione attraverso la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'attività scolastica e universitaria; la revisione della normativa in materia di appalti, con la previsione di strumenti in grado di valutare l'idoneità delle aziende in relazione all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, che diventa requisito indispensabile per accedere ad agevolazioni, finanziamenti e contributi di carattere pubblico. Allo stato attuale, inoltre, è stato predisposto lo schema di un decreto attuativo la cui adozione, ai sensi del disposto normativo, è prevista entro nove mesi In sostanza, si tratta di esercitare la delega entro il mese di maggio prossimo. È stata altresì predisposta una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di agevolare il coordinamento delle attività. della citata legge n. 123, che sono già in esercizio, vorrei ricordare alcuni dispositivi molto importanti. Il primo, all'articolo 3, è relativo al fatto che il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, promuove la cooperazione e il coordinamento per l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi. Tale documento è messo a disposizione delle rappresentanze sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare delle rappresentanze dei lavoratori alla sicurezza. sono stati avviati, già dall'anno 2007‑2008, progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state estese, con l'articolo 5, non solo all'edilizia, ma a tutti i settori imprenditoriali, le misure per contrastare il lavoro irregolare previste per il settore dell'edilizia all'articolo 36-*bis* del decreto Bersani nel caso in cui venga riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero quando si è in presenza di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro. Inoltre, viene prevista, ed è una forma profondamente innovativa, la possibilità di adottare il provvedimento interdittivo anche nel caso in cui vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. l'articolo 6 si è poi esteso l'obbligo del tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro per tutti i campi di attività, anche per quanto riguarda il lavoro autonomo, e all'articolo 8 è stato evidenziato che, per quanto riguarda le offerte degli appalti al massimo ribasso, il costo della sicurezza deve essere scorporato ed indicato in maniera specifica, così come specifica, così come che periodicamente, attraverso apposite tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si definiscono i livelli di retribuzione derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

l'articolo 9 sono state introdotte apposite sanzioni pecuniarie interdittive per le persone giuridiche i cui dirigenti siano responsabili di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro. Naturalmente, noi riteniamo che queste misure rappresentino un primo passo per la creazione di un meccanismo virtuoso che consenta il rispetto del lavoratore, in primo luogo, nella sua integrità psicofisica. Vorrei concludere rassicurando il Parlamento circa l'intenzione del Governo di proporre nell'immediato ulteriori misure. Per quello che ci riguarda, non si tratta di promulgare nuove leggi sulla tutela e sulla sicurezza del lavoro. Noi riteniamo che le leggi esistenti siano leggi avanzate,

Inoltre, abbiamo previsto, con la convocazione del prossimo Consiglio dei ministri, di portare all'approvazione i decreti del Presidente del Consiglio sulle attività di

è stata condotta di concerto tra il Ministero del lavoro e il Ministero della salute e che è stato stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo con le Regioni stesse

sono efficaci, il problema è della loro applicazione. Non solo, per un'efficace applicazione di queste leggi, è sicuramente necessario che nel nostro Paese si faccia strada una vera e propria cultura della sicurezza che deve coinvolgere tutti i soggetti interessati e che riguardi il sistema delle imprese. Bisogna passare ad una logica nella quale l'investimento in sicurezza non è soltanto un costo per l'impresa, ma una spesa utile al successo dell'impresa, alla qualità stessa dell'organizzazione del lavoro e alla valorizzazione delle risorse umane. devono essere valorizzati tutti quegli interventi di contrattazione sul luogo di lavoro che riguardano la prestazione lavorativa e la sicurezza dei lavoratori.

della nostra esperienza lavorativa e sicuramente un fattore, non soltanto negativo, ma anche doloroso, per le comunità coinvolte da questi continui lutti nel mondo del lavoro.

Chi ha vissuto - come ha fatto lui - i recenti giorni di Torino, avverte però tutta l'insufficienza delle parole di fronte al dramma di giovani vite spezzate in un inferno di fuoco. «Quella notte siamo andati a morire, non a lavorare» ha detto uno dei superstiti, esprimendo contemporaneamente paura, rabbia e rassegnazione; un legame tra lavoro e morte che pensavamo consegnato a tempi e Paesi lontani, limitato ad alcuni settori, vinto dalle tecnologie e dalle leggi e che è invece ancora in agguato, coglie un amico, un vicino di casa, spezza sorrisi e progetti. «Non si può morire per lavoro» hanno commentato in tanti a Torino, è assurdo. È proprio l'assurdità dei fatti della ThyssenKrupp che interroga la nostra responsabilità di legislatori, di amministratori, di uomini della politica e della cultura. Torino è ancora città operaia, un lavoro di fabbrica che allinea ambienti moderni e mansioni innovative con attività povere e pericolose, sovente in contraddizione con formazioni scolastiche ed umane di qualità. Vite in contrasto: quella difficile della quotidianità e quella delle aspirazioni e dei sogni, come la vita spezzata di uno dei ragazzi che, tra pochi giorni, si sarebbe dimesso dalla fabbrica per aprire un bar con la sua fidanzata. una realtà che forse abbiamo rimosso e abbiamo sostituito con l'idea di una società dai mille aggettivi che cancella dal proprio futuro gli spazi più difficili e meno interessanti. Ci avete dimenticato, hanno gridato i 30.000 del corteo di lunedì. Esprimevano proprio la rabbia di sentirsi abbandonati e messi da parte, non più protagonisti della vita della città e della sua storia. La prima lezione che dobbiamo imparare è proprio quella di rimettere in discussione l'analisi della società, di coniugare l'attenzione alla modernità con la tutela dei settori più deboli, di far sentire tutti protagonisti di un futuro che non è riservato soltanto a nuovi ceti e a nuove professioni. I morti della ThyssenKrupp, come quelli dei cantieri edili e dei troppi infortuni sul lavoro che segnano il nostro Paese, richiamano la giustizia e la responsabilità: due parole anch'esse gridate e invocate nella fabbrica e nelle assemblee, dal sindaco nel Consiglio comunale di Torino e dall'arcivescovo nella Chiesa della Consolata. Occorre sia fatta chiarezza sulle responsabilità, che emergano le negligenze e le trascuratezze. Lo stabilimento di Corso Regina stava per essere chiuso e trasferito: è legittimo chiedersi, dunque, se questa prospettiva non abbia allentato i sistemi di prevenzione ed abbassato la guardia della sicurezza. Risponderà la magistratura: se le accuse formulate in questi giorni dai lavoratori e dai sindacati si rivelassero anche soltanto in parte fondate, si configurerebbero responsabilità gravi, che dovranno essere perseguite con rigore; la domanda di giustizia non può rimanere senza risposta. In un'interrogazione, che ho presentato con i colleghi Bobba, Benvenuto e Negri, appena venuti a conoscenza dei fatti, ricordavo l'azione del Parlamento che ha approvato leggi importanti per la lotta contro gli infortuni sul lavoro. Ne ha diffusamente parlato il Ministro: abbiamo fatto la nostra parte, ma non vi è autocompiacimento in questa constatazione. Come ci ha ricordato il Ministro, occorre accelerare l'attuazione delle leggi, completare la preparazione del personale e creare le condizioni perché l'amministrazione pubblica sia in grado di prevenire e reprimere con efficacia e tempestività. La sicurezza del lavoro deve diventare parte integrante della cultura delle aziende, caratterizzarne l'organizzazione e modellarne i comportamenti. Si può fare, vi sono molti esempi virtuosi; non possiamo tollerare comportamenti differenti e negligenze interessate. Non si deve più morire di lavoro: è la prima condizione per la dignità della persona ed il presupposto per dare all'uomo il posto che gli spetta nell'organizzazione delle aziende e dell'attività economica. L'efficienza, il profitto, la capacità competitiva delle imprese sono fondamentali e anche la politica deve lavorare per accrescerle, ma non vi sono efficienza e competitività se non vi è la persona, se anche nell'attività lavorativa l'uomo non vede tutelato il suo primo diritto, quello alla vita. Con queste considerazioni, signor Presidente, concludo esprimendo la solidarietà del mio Gruppo ai familiari delle vittime e l'augurio di guarigione per i feriti*. (Applausi dai

Nel 1962, Dario Fo ed io eravamo conduttori di «Canzonissima» su RAI 1. Nell'ottava puntata avevamo pronto un brano sulle cosiddette morti bianche, problema già grave in quegli anni. I responsabili RAI censurarono il pezzo, così abbiamo scoperto che in Italia la gente non deve sapere che si muore sul lavoro. Ci siamo rifiutati di accettare il veto e abbiamo abbandonato la trasmissione, affrontando processi uno dietro l'altro e richieste di danni miliardari; per ben 16 anni siamo stati letteralmente cancellati da tutti i palinsesti televisivi. Oggi, dopo 45 anni, i *media* informano sulle quasi quotidiane vittime del lavoro: dal 2001 al 2007, si denunciano 8.376 morti, senza contare le innumerevoli malattie professionali che hanno colpito lavoratori (donne e uomini), la cui sopravvivenza è inesorabilmente segnata. Il nostro presidente del Consiglio Prodi ha commentato, tempo fa, che quei morti sono martiri del lavoro: no, Presidente, quei morti non sono martiri del lavoro, ma vittime uccise da atti criminali (lavoro nero e risparmio sulle impalcature di protezione). Cosa vale la vita di un immigrato clandestino? Cosa vale la vita di un lavoratore bianco in regola? Nulla: anch'egli può finire carbonizzato tra l'indifferenza generale; faccio presente che le mogli dei quattro operai deceduti bruciati a Torino sono disoccupate. Quello che vale è solo il profitto sulla pelle di chi è costretto a rischiare la vita ogni giorno per poter campare. Nel nostro Paese, milioni di persone vanno a lavorare tutti i giorni con il rischio di non tornare a casa, come se si recassero in un campo di battaglia. Gli infortuni sul lavoro costano alla comunità circa 50 miliardi di euro l'anno: se questa enorme somma fosse destinata alla sicurezza del lavoratore, oggi non saremmo ancora qui a fare i notai di questa triste conta dei caduti. Occorre urgentemente una struttura di controllo rapida e incorruttibile, che applichi una legge che colpisca severamente gli imprenditori disonesti, anche con la carcerazione, oltre a pesanti multe. Alcuni italiani si mettono in riga solo se li tocchi sui soldi; rispetto del loro prossimo ed onestà sono temi che non li riguardano; il loro cuore batte solo nel portafoglio e questo è vergognoso.

Signor Ministro, la sua analisi è stata certamente segnata da un'aritmetica drammatica, ma la tragedia delle acciaierie ThyssenKrupp era purtroppo, come molti sanno, una tragedia annunciata.

l'anticamera di una tragedia. Anche allora quelle fiamme si levarono altissime; anche allora l'incendio fu di vaste proporzioni e fu solo la fatalità, in quell'occasione, ad evitare altri feriti, altri morti ed altra disperazione. Da allora, a quanto sembra, il gruppo Thyssen ha deciso di non investire nemmeno sui più elementari sistemi di sicurezza e i rischi sono cresciuti, giorno dopo giorno, fino a sfociare in un dramma che si poteva, e probabilmente si doveva, evitare. Il resto è storia di ieri. Il corteo dei 30.000, una Torino operaia quasi dimenticata, spia della nuova paradossale decadenza del lavoro di fabbrica, il pianto di un padre che giustamente ha urlato al mondo la sua rabbia e il suo disprezzo verso i padroni, verso le istituzioni e verso il mondo. Oggi, il vero rischio resta l'oblio. Qualche riunione del Governo per orientare le iniziative e ribadire le leggi esistenti, il soprassalto di sdegno dell'opinione pubblica, destinato fatalmente a vaporizzarsi nei prossimi giorni, il sostegno alle famiglie, l'unica seria risposta di fronte al dramma delle vedove e degli orfani.

attraverso le sue nuove iniziative parlamentari. L'obbligo della politica è quello di restare vicino alla disperazione di chi è rimasto solo, anche quando le luci della cronaca si abbasseranno, anche quando questi morti verranno dimenticati. È questo il nostro dovere; proviamo tutti quanti a non dimenticare. Signor Presidente, colleghi, vorrei innanzitutto esprimere alle famiglie delle vittime di questo tragico incidente il mio più sentito cordoglio. In secondo luogo, vorrei rappresentare tutto il mio sconcerto nel constatare quanto ancora oggi si continui a morire sui luoghi di lavoro: quello di Torino, infatti, è solo l'ultimo tragico evento. Quattro vite strappate ai propri affetti solo per essere state al loro posto, come ogni giorno, al lavoro: un fatto intollerabile e inammissibile. Il Presidente del Consiglio ha parlato di una vera e propria emergenza nazionale: ogni anno un bollettino di guerra che con tragica puntualità miete migliaia di vittime, nei cantieri, nelle fabbriche come sulle strade. Ogni qual volta accadono simili episodi, ci si interroga sulla necessità di nuove regole per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Si tratta più probabilmente, già esistono, sia per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei lavoratori, sia per le sanzioni comminate alle aziende che non le rispettano. La carenza sta, piuttosto, nell'inadeguatezza e insufficienza dei controlli effettuati e nell'anomalia, tutta italiana, di non riuscire a far rispettare le norme vigenti. Non basta gridare con forza; dobbiamo operare a tutti i livelli affinché questo stato di cose non sia più accettato e muoverci per debellare questo flagello che non può più essere sopportato da una società civile. Bene ha fatto il Governo, durante il Consiglio dei ministri odierno, a decidere per l'accelerazione dei tempi per l'emanazione del testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi che ci auguriamo dunque possa trovare applicazione ben prima della naturale scadenza. Con riferimento al tragico incidente di Torino, invitiamo la magistratura competente ad accertare, nel più breve tempo possibile, responsabilità ed eventuali colpevoli, affinché la morte

per esprimere la nostra solidarietà ai parenti delle vittime, ma anche per evitare - lo dico con estrema franchezza ai rappresentanti del Governo la solita retorica che troppo spesso facciamo in queste occasioni. Credo ci siano due questioni che non possono sfuggire di fronte alla tragedia di Torino. Una

in una fabbrica di grandi dimensioni, quindi, con tutti quei criteri che dovrebbero normalmente garantire le condizioni di sicurezza (la rappresentanza sindacale ufficiale,

nel Paese. Senz'altro ci può essere un problema di aggiornamento e di perfezionamento delle norme in vigore; in assoluto, è chiaro che qualsiasi legge può essere perfettibile, ma mai, come in questo caso - se ho ben capito, e del resto anche la mia esperienza di Governo mi porta mi porta alla medesima conclusione - c'è un problema che riguarda i controlli e le verifiche del rispetto delle disposizioni, che purtroppo siamo stati abituati, per troppo tempo, a considerare soltanto un fenomeno che attiene al livello della sottoccupazione, laddove esiste, cioè, trascuratezza del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro previste del nostro Paese o una endemica situazione di lavoro sottoccupato o in nero,

a tutti i livelli: riguarda le rappresentanze del lavoro, ma anche la rappresentanza dell'industria, perché non scatti quel meccanismo

alcuni mesi fa, abbiamo discusso questo tema ed è venuto fuori che l'INAIL intendeva ridurre le proprie tabelle su invalidità e morti sul lavoro. Mi auguro che il Governo sia intervenuto e l'INAIL abbia cambiato idea. Sento dire che alla Camera verrà utilizzato il tesoretto dell'INAIL. Mi pare, anche per le parole del Ministro, che nella prevenzione e nel controllo ci siano delle maglie molto larghe e dei buchi di una certa consistenza; quindi, non è cosa molto positiva il tesoretto che l'INAIL

è l'ultimo problema che si pongono e vi è un rapporto incredibile tra numero di aziende e numero di tecnici a disposizione. Ultima questione: leggo oggi sui giornali che il ministro Turco afferma che il modello è l'ILVA di Taranto.

le istituzioni e le forze politiche pensarono bene di aumentare di 60 volte il limite del PCB e di 1.000 volte il limite fissato dalla normativa europea per la diossina.

conti il minuto di raccoglimento per chi muore sul lavoro, ma si comincino a contare anche le decine e decine di morti causate dai gas combusti, come scientificamente dimostrato da studi internazionali, di fronte alle quali ci vogliono chiudere gli occhi.

siamo sopraffatti dalla certezza che non basta più la pur sentita solidarietà con le famiglie delle vittime; non basta più puntare transitoriamente i riflettori sull'autentica emergenza costituita dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, né basta più farlo ritualmente dopo ogni sciagura. Questo è ormai il tempo delle risposte concrete, degli interventi puntuali e rigorosi; è il tempo dei fatti, innanzitutto per rendere giustizia ai familiari delle vittime. Le inadempienze ed i buchi neri nel sistema di prevenzione alla ThyssenKrupp rimandano a gravissime responsabilità che vanno individuate e colpite, ma non c'è solo questo: sono la rabbia e il senso di abbandono che vivono i lavoratori, che denunciano un corto circuito di enorme gravità tra il lavoro salariato, la politica e, financo, il sindacato. Siamo d'accordo con chi sostiene che la politica tende a non vedere più ciò che non le piace, che gli operai non sono più di moda e che c'è il rischio che nessuno si occupi più della loro ordinaria infelicità, dei loro problemi di ogni giorno. C'è una distanza eccessiva tra il linguaggio e gli argomenti della politica e la dura realtà del lavoro operaio. Occorre, invece, intanto, dare continuità ad una legislazione, pur positiva, che richiede l'attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 123 del 3 agosto 2007, a partire dalla tempestività dei provvedimenti (nove mesi sono troppi!), fino alla razionalizzazione ed al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza per garantire la capillarità e la tempestività

Occorre far presto, occorre cogliere il costante monito del presidente Napolitano sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché ne va della credibilità dello Stato.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, noi della Sinistra riteniamo che non sia possibile comprendere la tragedia di Torino ed il dramma, che giorno dopo giorno si ripete, delle morti e degli incidenti sul lavoro, se non si guarda negli occhi il degrado della condizione lavorativa esistente oggi in Italia. Se non si parte da qui non si reagisce nel modo giusto, serve una reazione forte, determinata e tempestiva. Il Ministro ci ha detto che non servono misure di emergenza; può darsi, ma è certo che serve una svolta. Sarei insincero se dicessi che nelle parole del Ministro abbiamo avvertito la necessità e l'urgenza di questa svolta. Chiediamo che si faccia di più e di meglio e che si inverta la rotta su molti punti, a cominciare dalla legislazione sul lavoro. Il Governo dice che non serve un decreto‑legge. Spero che questo giudizio non nasca dal fatto che questa volta la responsabilità dell'omicidio non ricade su un emarginato, ma su una grande impresa; non ricade su zingari, ma su tedeschi di pura razza ariana. Trovo estremamente grave l'arroganza che la ThyssenKrupp sta manifestando fino al punto di rifiutare oggi di incontrare la delegazione della Commissione per gli infortuni sul lavoro del Senato. Chiedo al presidente Marini di attivarsi per contestare questo atteggiamento. O credono di stare nella Namibia di cento anni fa! Decreto-legge o no, chiediamo al Governo un cambio di passo anzitutto sulle grandi questioni delle condizioni del lavoro e dei lavoratori. La tragedia di Torino sta svelando al Paese l'esistenza di una grande questione: la questione operaia. Come ricordava il senatore Montalbano della questione di milioni di lavoratrici e lavoratori i cui salari si riducono anno dopo anno, che rischiano di perdere il posto di lavoro da un giorno all'altro, che se sono giovani hanno contratti di lavoro precari, senza sapere se potranno ancora lavorare la settimana o il mese dopo, e che se sono meno giovani non solo devono mantenere una famiglia con poche centinaia di euro al mese, ma vengono anche additati al Paese come i privilegiati, i garantiti, coloro che tolgono il pane dalla bocca ai giovani. I morti e i feriti di Torino sono gli stessi operai che avevano lottato contro la chiusura della fabbrica per non rimanere disoccupati; sono compagni di sventura di quelle migliaia e migliaia di vivi che ancora oggi possono essere costretti, se una grande multinazionale lo esige, a lavorare dodici ore al giorno, se vogliono continuare ad avere quel dannato posto di lavoro per consentire almeno di non passare un Natale di fame. Questo accade non in Asia, ma in Italia, a Torino, grande città operaia. Questo accade nello stabilimento di una delle grandi e moderne multinazionali il cui comportamento insensibile e arrogante è la migliore prova che per costringere le grandi imprese a rispettare i loro dipendenti servono leggi severe e controlli intransigenti; servono misure che quando sono violate le colpiscano nel cuore, che è il portafoglio; serve una grande determinazione da parte della politica e delle istituzioni, che hanno il compito di difendere coloro che nella società dei brutali rapporti di forza della globalizzazione neoliberista sono altrimenti abbandonati a se stessi. Ripeto: stiamo parlando non di lavoratori sfruttati in qualche Paese asiatico, ma di operai, cittadini di una Repubblica fondata sul lavoro, ai quali la Costituzione promette diritti che le leggi della Repubblica non riescono a garantire e che la politica non riesce a fare valere. I cantori della modernità avevano descritto negli anni del liberismo trionfante - che qualche tardo epigono continua ancora a magnificare a magnificare - una nuova economia fondata sui beni immateriali e una società nella quale, affidandosi alla mano invisibile e provvidenziale del mercato e del profitto, ci sarebbero stati benessere e felicità per tutti. La realtà dei fatti ci dice, invece, che così non è; ci dice che la questione operaia è più aperta che mai. Vi sono milioni di operai la cui attività produttiva seria e professionale è decisiva per il benessere di tutti; tutti; sono diventati marginali non perché il loro ruolo sia tale, ma perché così vuole e così esige la cultura dominante della società in cui viviamo, se è vero che il maggior telegiornale della televisione di Stato ha aperto la sera della tragedia il notiziario con un'opera lirica seguita da alcune irruenti dichiarazioni dei politici di turno e, solo a quel punto, ha ritenuto giusto dare notizia di quanto accaduto. Gli operai guadagnano sempre meno, le condizioni di lavoro in fabbrica sono sempre peggiori, la mobilità sociale è un ricordo del passato perché è sempre più difficile per il figlio di un operaio

Se non si parte da qui non si comprende la terribile verità delle morti sul lavoro. La politica deve riproporre la questione operaia al centro della sua agenda, non con le chiacchiere, né con la retorica della commozione che dura quarantotto ore, ma dando il segno di comprendere quello che accade e di voler agire per cambiare lo stato di cose esistente. La sinistra unita pone questo tema questo tema e lo fa su due livelli, entrambi decisivi: il primo riguarda specificamente la questione sicurezza, il secondo la condizione salariale e i diritti dei lavoratori in fabbrica, due aspetti strettamente collegati. La nuova legge sulla sicurezza è stata approvata ad agosto; il Governo aveva a disposizione nove mesi di tempo: sono passati più di quattro mesi e ancora le bozze di decreto non sono state consegnate alle parti sociali. A quanto si sa, c'è stato un defatigante rimpallo tra gli uffici del Ministero del lavoro, quello della sanità e le Regioni. Ora si recuperi il tempo perduto. Al riguardo c'è da tempo un'evidente questione istituzionale aperta e legata al moltiplicarsi delle competenze che determina inefficacia e scarico di responsabilità. Fra le tante riforme istituzionali di cui si parla ce ne è una urgente: modificare l'errata scelta compiuta nel Titolo V della Costituzione, che affida la legislazione concorrente in materia di sicurezza del lavoro allo Stato e alle Regioni. Ancora oggi le ASL non sono in grado di fare la loro parte e le Regioni non si occupano a sufficienza di questi temi. Ancora questa mattina la responsabile della ASL di Torino non ha risposto ai quesiti che le sono stati posti dalla Commissione presieduta dal senatore Tofani. Ci sia, invece, un unico centro di responsabilità politica e istituzionale affidato al Parlamento e al Governo nazionale. Questo, naturalmente, non può essere un alibi per non stringere i tempi delle decisioni: ogni giorno che passa senza interventi seri e concreti per prevenire e ridurre il più possibile gli omicidi bianchi è un giorno perduto. È dunque opportuno fare poche cose, ma concrete e urgenti. Il Governo richiami le imprese al rispetto della normativa esistente; il Governo emani al più presto i decreti delegati previsti dalla legge di agosto; il Governo si faccia subito parte attiva per incidere sulle condizioni di lavoro in fabbrica.

È uno scandalo! Non deve essere più possibile quello che è accaduto a Torino, dove gli operai sono stati sottoposti al ricatto tra lavorare dodici ore in una sola giornata o restare disoccupati.

«Se otto ore vi sembran poche» cantavano le nonne dei morti di Torino. In secondo luogo, il Governo si attivi per chiedere alle imprese i rinnovi dei contratti di lavoro privati aperti, oltre che per rinnovare tempestivamente il contratto del pubblico impiego. Concertazione non vuol dire attendere passivamente che le parti si mettano d'accordo; a partire dal luglio 1993 il Governo è parte istituzionale e garante anche del rinnovo dei contratti privati e non può continuare ad assistere passivamente all'ostruzionismo confindustriale di fronte a contratti nazionali che da anni non vengono rinnovati e che riguardano milioni di lavoratori: i metalmeccanici, i giornalisti, le commesse, le addette alle pulizie. Tutti ormai dicono che i salari sono troppo bassi, che senza crescita salariale il Paese intero non cresce. Lasciamo perdere prese in giro come il *Mister* prezzi. prezzi. Se vogliamo reagire alla perdita di potere d'acquisto dei salari la prima misura è rappresentata da nuovi contratti che prevedano stipendi e salari più dignitosi. Il Governo esprima con chiarezza e fermezza il suo giudizio e il suo punto di vista: non c'è posto per Ponzio Pilato davanti al diritto a un trattamento economico dignitoso previsto dalla nostra Costituzione. Il dramma degli infortuni dà anche una ragione in più per combattere le condizioni di precarietà nei posti di lavoro. Quanto previsto nel protocollo anche a questo riguardo è davvero troppo poco; certamente non ci basta. Cito solo un dato. Un ruolo centrale nel sistema della tutela contro gli infortuni è assegnato ai rappresentanti sindacali per la sicurezza. Ma come si può pretendere che questi lavoratori possano contestare le inefficienze, le insufficienze, le violazioni delle leggi sul lavoro se sanno che dipende dall'arbitrio della controparte se potranno continuare o no a conservare il posto di lavoro? Bisogna cambiare la legge n. 30 del 2003, bisogna contrastare il precariato, non basta dire - come pure è giusto - che dalle mansioni pericolose vanno esclusi i precari. E ancora, c'è una responsabilità sociale dell'impresa e, in particolare, della grande impresa da affermare nelle leggi dello Stato e non solo nei convegni di Confindustria. L'Italia ha una legislazione che prevede la responsabilità civile e penale della persona giuridica. Bisogna utilizzarla di più e meglio, bisogna prevedere la responsabilità civile e penale della persona giuridica anche nelle ipotesi di *outsourcing* e nell'intera catena delle attività lavorative che fanno capo all'impresa madre; bisogna invertire la logica della convenienza economica, la sanzione pecuniaria deve essere tale che nei costi d'impresa non sia più economicamente conveniente, come invece è oggi, violare le leggi che tutelano il diritto alla vita e alla salute dei dipendenti. Come si vede, non formuliamo richieste né ideologiche, né massimaliste. Chiediamo misure concrete, non solo perfettamente compatibili con la logica produttiva, non solo tali da ridare al lavoro il valore sociale e la dignità perduti, come è necessario e giusto in sé, ma come è anche indispensabile per dare all'Italia una competitività globale che sia alta, di sistema. O credete davvero che possiamo competere con l'economia asiatica nel ribasso dei salari, dei diritti, della sicurezza del lavoro? Misure concrete, misure serie, misure urgenti. Queste misure è giusto esigerle con grande determinazione. Quando chiediamo al presidente Prodi nuova determinazione, nuovo impegno se vuole rilanciare l'azione di Governo chiediamo anzitutto - e abbiamo il diritto e il dovere di chiederlo e di pretenderlo - che si dia alla questione operaia e alla questione sociale aperte in Italia la centralità che meritano. Altrimenti gli operai avranno davvero ragione di fischiare, di fischiarci tutti, di fischiare una politica che si dilania sulla legge elettorale, che minaccia sfracelli per questo e per quello e che davanti ai morti del lavoro è capace solo di parole e di presenziare solennemente ai funerali. L'unità della sinistra, la Sinistra l'Arcobaleno nata domenica a Roma, che mi ha fatto l'onore di chiedermi di parlare a nome di tutti i Gruppi parlamentari che la rappresentano in questo ramo del Parlamento, la sinistra unita nasce anche per questo. Forse nasce soprattutto per questo. Abbiamo preso e prendiamo un impegno per onorare chi è morto e per tutelare chi è vivo, l'impegno di ripristinare la dignità del lavoro che è dignità dei diritti e dignità del reddito. Questo impegno noi lo onoreremo fino in fondo.

ringrazio il ministro Ferrero per la sua relazione molto completa che ci consente di andare oltre la cronaca e di guardare lontano. Ai giorni del dolore e della rabbia, infatti, dobbiamo ora impegnarci a far seguire i giorni della riflessione e delle analisi; se necessario, dei giudizi e dei processi. Ma prima è giusto rivolgere ancora una parola di cordoglio, senza ritualità, alle famiglie delle vittime, ma anche una parola di solidarietà, di augurio ai feriti affinché possano ristabilirsi in fretta e possano soprattutto dimenticare, con l'aiuto del tempo, il ricordo di quell'inferno terribile al quale sono scampati. Dopo i processi di piazza, che per bocca dei 30.000 dimostranti di Torino,

per evitare che tutti paghino per tutti e che qualcuno magari riesca a farla franca. Eventi così gravi, sentimenti così disperati non possono avere colore politico, né distinzione di ruoli. Per questo è giusto aver sigillato la fabbrica al fine di agevolare gli accertamenti e le responsabilità interne, ma è altrettanto opportuno verificare le corresponsabilità esterne o indotte di chi doveva prevedere, di chi doveva controllare e non lo ha fatto. Ancora più utile ora è far tesoro di questa tragica lezione e guardarci attorno, guardare a tutte le realtà produttive in cui il processo lavorativo pone le persone a stretto contatto quotidiano con il pericolo. Spesso all'eventualità estrema, anche alla più tragica, si fa quasi l'abitudine, si abbassa la guardia e quindi si resta vittime dell'imprevisto: è a quel punto che l'apparato aziendale, ma non solo, anche quello sindacale, debbono intervenire con richiami efficaci e con iniziative opportune. Le campagne per l'uso del casco, dei guanti, degli occhiali e così via non possono più occorre intervenire sugli orari di lavoro e sui tempi di recupero, per evitare che il superaffaticamento abbassi l'attenzione, faccia abbassare la guardia. Occorre anche, anzi soprattutto, però, intervenire sui salari per mantenerli competitivi con l'aumento del costo della vita ed evitare che la perdita del potere d'acquisto costringa operai ed impiegati ad intensificare il ricorso al lavoro straordinario o peggio, come già è stato osservato, al lavoro nero. Di questa sconfitta del salario nei confronti del mercato deve farsi carico proprio il Governo con riforme vere, non con interventi demagogici come gli esigui aumenti salariali, oppure l'impercettibile riduzione della pressione fiscale sulle famiglie. Da Confindustria e anche da altre organizzazioni imprenditoriali, proprio in questi giorni, stanno giungendo segnali diversi, segnali coraggiosi, nella direzione di una rigorosa pulizia interna, di una responsabilità a trecentosessanta gradi nell'impegno per la sicurezza; ma si respira anche una seria volontà di mettere mano alle riforme di base. Tocca ai sindacati ora fornire risposte adeguate, cercando magari parole nuove, parole diverse rispetto a quelle che hanno reso difficile, in passato, il dialogo e soprattutto hanno reso impraticabile il percorso delle intese. L'ondata di dolore che la tragedia di Torino ha sollevato ha risvegliato molte coscienze e ha fatto comprendere che un evento luttuoso è il segnale di un allarme più generale che coinvolge un intero sistema, un sistema che non funziona e non solo di un apparato a rischio: chi ha l'onere e l'onore di governare ha anche il dovere di dimostrare di saper cogliere tali segnali per trasformarli in azioni coerenti ed efficaci ed evitare che simili lutti, che appartengono a tutti noi, si ripetano, per non ridurre la nostra reazione, la nostra responsabilità, ad un dibattito come questo. "Ognuno deve fare la sua parte" ha detto, poco fa, il presidente Marini. Ebbene, la nostra parte è di stimolare il Governo ad azioni concrete, affinché tutti gli interrogativi abbiano una risposta ed ogni responsabilità una sanzione, senza sconti per nessuno. Ma la nostra parte di rappresentanti dei cittadini è anche quella di stringerci attorno alle famiglie delle vittime per non lasciarle sole con il loro dolore ed i loro problemi e garantire loro che l'ondata di solidarietà non sfumerà, non scemerà con i giorni ed i mesi, finché un nuovo lutto consegni un altro dramma così grande, o anche di più, al triste catalogo delle sciagure quotidiane del nostro Paese, insieme alle molte altre, purtroppo, del passato e in attesa

Non cogliere questa lezione generale, questo respiro umano prima ancora che politico, non avvertire il peso di questa responsabilità morale renderebbe ipocrite le nostre parole di oggi e sarebbe un po' come fare morire due volte gli sventurati operai di Torino, eroi moderni su un fronte di pace in cui, tuttavia, si continua a morire, proprio come in una guerra senza fine, mai dichiarata, ma presente, ovunque, ogni giorno.

altre, perché è abbastanza stucchevole, anche se la politica ha le sue liturgie, fare questo tipo di interventi, di dibattiti subito dopo una tragedia, tutti a dimenticarsene presto, in attesa di quella successiva. Vorrei iniziare, prima di tutto, con un pensiero veramente deferente e di vera vicinanza,

In tal senso credo che lo Stato potrebbe fare qualcosa di estremamente tangibile. In anni in cui si sperpera veramente il denaro pubblico

la pubblica amministrazione non dovrebbe avere nessuna difficoltà ad avere un fondo proprio di risarcimento immediato per le famiglie delle vittime sul lavoro, indipendentemente da tutto il resto, che garantisca, per lo meno nel dolore e nella tragedia, la tranquillità economica a chi resta dopo questi gravissimi fatti. Dopodiché, signor Ministro, sia per il suo intervento, che mi aspettavo un pochino più dettagliato sull'avvenimento e che, in realtà, è stato alla fine uno *spot* elettorale di quanto ha fatto pretende di aver fatto il Governo in questi diciotto mesi, sia per gli interventi dei colleghi della maggioranza che mi hanno preceduto e che hanno approfittato di questa situazione per fare una sorta di manifesto

argomenti, su cui forse tutti insieme dovremmo riflettere: innanzitutto la questione della legislazione. Si continua ad insistere sui provvedimenti legislativi. Ricordo che l'Italia ha una

con una legislazione anche molto più severa, comunque non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Visto che tutti i colleghi della sinistra sono intervenuti, invece, ribadendo i concetti storici di sempre che conosciamo tutti, vorrei fare una riflessione su questo. Torino, come giustamente è stato detto, non è una città del profondo Sud italiano o del profondo Sud del mondo: è una città dove la sinistra governa da sempre, dove la tradizione operaia è fortissima e la presenza sindacale è altrettanto forte. Non mi si venga a dire che i sindacati della ThyssenKrupp di sudditanza psicologica nei confronti della proprietà, perché questo veramente non lo crederebbe nessuno. Quindi, c'è qualcos'altro che non va. Anche dove la cultura della fabbrica e del lavoro teoricamente non dovrebbero mancare, ugualmente si è arrivati ad una situazione

i controlli, probabilmente superflui, e che sarà rispettato esclusivamente da quelle aziende che già oggi rispettano la legge. legge. Anche qui non si può fare di tutta l'erba un fascio, perché citare un dato numerico e basta, oltre a non essere assolutamente indicativo della realtà del Paese, è anche fuorviante circa la direzione da prendere per cercare di risolvere il problema.

che ovviamente, se sono assolutamente importanti dal punto di vista della gravità del fatto, è evidente che non vengono coperte dal premio pagato dalle aziende all'INAIL, perché il problema riguarda il controllo stradale o la sicurezza delle strade. degli incidenti, per la gran parte, avviene purtroppo nei cantieri edili, dove effettivamente è più diffusa

sui contenuti e non sulle questioni inutilmente polemiche della politica, devo dire che qualche provvedimento, di quelli più semplici fatti da questo Governo, è assolutamente da condividere; penso, ad esempio, a quello dell'assunzione il giorno prima dell'inizio del lavoro:

di rispetto e stima reciproca tra l'imprenditore e i collaboratori, ma anche - se vi piace di più, visto che siete cultori del materialismo - perché semplicemente non conviene economicamente già oggi.

dove forse - e qui sì bisogna fare qualche altra riflessione - la spersonalizzazione del lavoro e del rapporto tra le persone porta a situazioni come quella di Torino. di Torino. Tutte le altre riflessioni che si sono fatte sul lavoro precario, sul lavoro instabile, e tutto il resto lasciano il tempo che trovano, perché non in tutti i Paesi c'è una legislazione come quella italiana. non esiste il contratto a tempo indeterminato come lo intendiamo noi, ma dove c'è la cultura del lavoro queste cose non succedono perché le persone sono comunque attrezzate mentalmente e culturalmente per il lavoro che stanno facendo. Se ho ancora qualche istante, signor Presidente, vorrei fare un'altra riflessione. Colleghi, usciamo dalla retorica: non si deve morire di lavoro, è giusto, ma in un Paese civile non si dovrebbe morire di tante altre cose.

per via dei criminali usciti di galera; alle persone ubriache per la strada che ammazzano i ragazzi, ai magistrati che rilasciano liberi criminali impenitenti i quali poi si mettono al volante e ammazzano persone: tutto

O qui si vuole tornare ad essere un Paese dove la legalità esiste dappertutto, a partire dai luoghi di lavoro, oppure è inutile oggi venire qui a celebrare questa liturgia, in attesa della prossima. Un'ultima considerazione, di carattere numerico ed economico.

che proprio nei Paesi dove non c'è il profitto capitalista, per esempio nella Cina rossa, tutti gli anni muoiono 7.000-8.000 persone nelle sole miniere di Stato, senza che nessuno dica nulla. Ragioniamo anche sul nostro Paese: in Italia siamo 60 milioni di persone, di questi lavorano solo 23

da tutti coloro che sistemiamo negli enti, a centinaia di migliaia di euro l'anno pagati dalle tasse di questi 2 milioni di lavoratori, dovremmo farla. Cominciamo tutti a rinunciare a qualcosa, a rispettare il mondo del lavoro a partire dai dipendenti, dagli operai, dalle fabbriche, e a dare al mondo del lavoro i mezzi per produrre ricchezza in maniera sicura. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto, a nome dell'UDC, esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime di Torino. È assurdo che ancora oggi così tanti lavoratori mettano a rischio la propria vita semplicemente andando a lavorare tutti i giorni, e che la rete di sicurezza sia ancora così carente da causare incidenti mortali. Di fronte a questo non ci possono essere divisioni politiche o visioni di parte. L'obiettivo deve essere comune: salvaguardare la sicurezza delle persone sul luogo di lavoro evitando che esso si trasformi in una trappola mortale. Da troppo tempo, purtroppo, assistiamo ad episodi del genere senza che nulla di significativo sia cambiato, e crediamo che non sia responsabile da parte della politica rimandare la soluzione del problema, perdendosi in discussioni inutili e sterili. Senatore Salvi, è un argomento troppo serio e delicato perché diventi terreno di scontro o di strumentalizzazione a fini politici e demagogici. Ecco perché invito tutti ad astenersi dalla facile tentazione di addossare colpe o accuse all'avversario e di tentare seriamente di risolvere il problema. soluzione non deriva dall'inasprimento delle misure legislative e sanzionatorie né dalla condanna senza appello, e direi senza neanche processo, del mondo imprenditoriale, perché non si può dimenticare che la grande maggioranza delle aziende rispetta rigorosamente le regole in materia di sicurezza. Sarebbe sbagliato gettare la croce addosso all'intero mondo imprenditoriale, indicandolo disponibile a sacrificare la vita umana sull'altare della competitività e del profitto. Dietro ad ognuno di questi incidenti ci sono negligenze, talvolta imprudenze, spesso semplici fatalità. Situazioni diverse e responsabilità diffuse che investono in modo graduale, ma non per questo meno grave, tutti gli operatori economici e sociali che gravitano intorno al lavoro. Oggi non serve sciorinare statistiche e numeri, anche per rispetto delle persone morte, perché sarebbe un inutile esercizio retorico. Andrebbe piuttosto spiegato perché, non più di sei mesi fa, questa stessa Assemblea ha votato senza battere ciglio la proroga di nove mesi per l'esercizio della delega in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Prendo atto con soddisfazione che oggi lei, signor Ministro, ritiene necessaria un'accelerazione dell'attuazione della delega. Forse fino ad oggi non si riteneva abbastanza urgente intervenire realmente nella sostanza del problema, ma utilizzarlo per vuoti dibattiti mediatici. Oppure nella vostra agenda politica era più importante occuparsi della sicurezza urbana e delle «terribili discriminazioni» nei confronti delle identità di genere, sulle quali avete persino rischiato di far cadere quel Governo delegato a legiferare sul tema del lavoro? La delega, peraltro, risulta improntata, per motivi ideologici, ad una logica punitiva ed un aumento delle sanzioni, che, come ben sappiamo, hanno da tempo esaurito la loro efficacia deterrente. Per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro serve a poco continuare ad invocare nuove leggi. Signor Ministro, concordo con lei: quelle già esistenti sono assai avanzate e, semmai, a mio avviso, peccano di eccessi burocratici. Allo stesso tempo è vano rincorrere la retorica dei controlli come panacea di ogni male. Proprio in tema di controlli, non abbiamo bisogno di nuove norme, ma di conferire al sistema sia maggiore collegialità che maggior coordinamento tra gli enti preposti, di una semplificazione di tutti quegli oneri amministrativi che spesso assediano gli imprenditori, senza peraltro garantire i lavoratori. In questi anni di applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 dovrebbe essere diventato palese a tutti che né gli eccessi burocratici, né quelli sanzionatori, possono garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o contribuire a proteggere i lavoratori. Dovrebbe essere ormai maturata la consapevolezza che il maggior rispetto della normativa vigente si possa fondare non solo sul consueto meccanismo sanzionatorio, la cui effettività peraltro risente di una cronica mancanza di risorse e mezzi, ma anche sulla predisposizione di un percorso che sia capace di venire incontro alle carenze di formazione, informazione e prevenzione. Sono d'accordo con lei, signor Ministro, c'è bisogno di cultura della sicurezza: servono giovani preparati e consapevoli dei rischi che dovranno affrontare e delle responsabilità che dovranno sostenere, siano essi in futuro lavoratori o imprenditori. Occorre ripensare integralmente un sistema dove entrambi saranno chiamati a condividere le risposte ai problemi che necessariamente si presenteranno e dovranno essere affrontati senza dannose contrapposizioni e superficiali rivendicazioni. La soluzione del problema, in conclusione, non sta nel creare un sistema di regole complicato, in cui è difficile districarsi, o nell'assumere in massa ispettori, creando un clima di terrore. Occorre piuttosto rendere effettivi ed efficaci i controlli, soprattutto dove si sa benissimo che esistono ampie sacche di lavoro nero, in un rapporto essenziale di coinvolgimento di tutte le parti sociali. Il Governo non utilizzi come uno *slogan* l'alibi della scarsità di risorse, perché nell'ambito delle leggi finanziarie si poteva, e si potrebbe ancora, destinare strumenti finanziari ed umani al problema della sicurezza sul lavoro, evitando i tanti sprechi e gli interventi inutili e clientelari. Il problema investe l'etica della politica: se tutti questi morti non suscitano indignazione e non inducono tutti, dico tutti, ad un cambiamento nei comportamenti, saranno state morti inutili. Tutti, politici, imprenditori e sindacati, sono quindi chiamati ad un'assunzione di responsabilità e ad affrontare il tema del lavoro non con visioni parziali, ma in modo sistematico, coniugando problematiche salariali, forme contrattuali e sicurezza. Questo perché, anche se cambia l'economia, se cambiano le relazioni industriali e le tipologie di lavoro e di contratto, ciò che non deve mai essere perso di vista è il valore della persona e della vita. *(Applausi

Signor Presidente, colleghi senatori, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha lavorato attentamente, nel corso di questa legislatura, sui problemi connessi alla sicurezza; non vi è dubbio,

qualche notizia che ci arriva da quella città, dove la nostra Commissione è impegnata a svolgere le audizioni e a visitare il luogo del disastro. In ogni caso, se soltanto fossero confermate le prime dichiarazioni provenienti dai superstiti di questa immane tragedia, ci troveremmo di fronte ad un fallimento ben più ampio di quello che si registra per un'inadempienza dal punto di vista della sicurezza. Signor Ministro, se quegli estintori fossero stati davvero scarichi, ci troveremmo di fronte ad un problema gigantesco, che coinvolgerebbe, evidentemente, non soltanto l'azienda, ma anche le autorità che avrebbero dovuto svolgere i controlli e - perché no? - anche, forse, di fronte ad un'attenzione non propriamente rispetto ai problemi che vengono normalmente posti, come lei sa, in una semestrale, persino da parte delle forze sociali. Il fatto che un settore maturo e, se vogliamo, obsoleto,

che a tutta questa situazione si possa rispondere semplicemente affermando che non occorrono provvedimenti straordinari: probabilmente, signor Ministro, occorrono straordinari salti di maturità politica e culturale da parte dell'intera classe dirigente.

sia un primo elemento di riflessione: certo, occorre, sì, una legge straordinaria, costituzionale, per ricomporre e riportare ad unità quella frammentazione, perché evidentemente i controlli non funzionano. Da Torino, signor Ministro, apprendiamo una vicenda sconcertante: l'attesa, a mio avviso francamente inaccettabile, sul piano del rispetto istituzionale reciproco, della nostra Commissione d'inchiesta davanti ai cancelli per oltre un'ora, prima che le venisse concesso di accedere al luogo del disastro. Oltre a ciò, ci vengono notizie importanti già dalle audizioni: il procuratore capo, il dottor Maddalena, ha già parlato esplicitamente di controlli insufficienti in generale; ha sottolineato, inoltre, l'insufficienza delle ispezioni da parte delle ASL. A Torino, signor Ministro, il dirigente delle ASL, che in audizione avrebbe dovuto fornire qualche risposta rispetto a tali insufficienze,

non risolviamo il problema della sicurezza assumendo più ispettori, come non risolveremmo quello della sanità assumendo più infermieri: certamente, è meglio averne di più che di meno, ma occorre una razionalizzazione di questi strumenti, che al momento manca. Mi permetta poi di uscire dal contingente di questa tragedia, che pure segna questo dibattito e segna anche un momento importante di riflessione dell'intero Paese su questi temi. Ma guardi che, al di là di questa tragedia, ben oltre si consuma ormai sotto i nostri occhi, proprio per una carenza culturale presente nel Paese; vi è un problema di rischio costante che attraversa il processo del lavoro, persino dal momento dell'intermediazione. Guardi che Roma, la capitale d'Italia, oggi assomiglia a quei Paesi - lo dico a lei che, per sua estrazione, può capirmi meglio di altri - che venivano descritti dai grandi intellettuali della sinistra, su "Rinascita", come Paesi privi di democrazia, perché c'era il caporalato. Ebbene, signor Ministro, faccia una volta ciò che ho fatto io, ma non perché sia tenuto a farlo; passi alle passi alle ore 6 di mattina a Ponte Milvio e vedrà che in questa città, sotto i nostri occhi, a qualche chilometro da quest'Aula, ogni mattina passano i furgoni e reclutano personale che va certamente a svolgere lavoro illegalmente. Noi siamo andati ad intervistare queste persone e ci raccontano di infortuni che non hanno mai denunciato; ci raccontano di come qualche amico medico fa nascondere loro le contusioni e poi tornano a lavorare quando si sono ripresi. Quando uno di questi incidenti sarà più grave, noi saremo in quest'Aula e non potremo cadere dalle nuvole, signor Ministro, perché questa è la realtà della capitale d'Italia: 1400 persone, ogni mattina,

Allora, le tragedie annunciate potranno concludersi soltanto quando la nostra classe politica riuscirà a superare l'antico inciampo di pensare che su queste questioni conta il richiamo retorico più tonitruante in quel momento o conta il richiamo meramente di classe. C'è un problema più serio; c'è un problema di cultura del lavoro che certamente si deve fare strada e che certamente deve entrare nel DNA di un nuovo corso, che manca. In questo momento, questa privazione offende certamente i ceti operai; domani offenderà l'immigrazione clandestina; dopodomani forse potremo scoprire che in qualche infinitesimale subappalto, anche qui, anche a Roma - come appare proprio oggi sui giornali anche negli appalti normali e nei lavori normali che si effettuano sui binari delle ferrovie, l'incidente è in agguato. Bene, facciamo questa riflessione. Quest'Aula su questo non le è pregiudizialmente né amica né nemica; non è un tema su cui l'Aula del Senato si divide per colori o per parti politiche. L'abbiamo dimostrato molte volte, e le ha ricordate quasi tutte il presidente Marini. L'ultima occasione la voglio ricordare io, ed è stato durante la finanziaria, quando è passato un emendamento, che aveva come primo firmatario il nostro collega Oreste Tofani, che ha esteso il diritto di collocamento obbligatorio agli orfani o, in alternativa, ai coniugi superstiti di coloro che sono stati vittime di incidenti sul lavoro. Dunque, signor Ministro, come vede, c'è una grande attenzione. Il suddetto emendamento, se non ricordo male, fu approvato C'è una grande attenzione e uno spirito costruttivo sano nel Parlamento rispetto a tali questioni. Abbiamo bisogno di un Esecutivo che raccolga questi spunti e che non stia ad indugiare su una serie di rituali e anche sulla mera rappresentazione statistica di un fenomeno che, per moltissime ragioni, quando tocca una delle più importanti città industriali italiane, nelle condizioni in cui è accaduto questo incidente e nelle modalità che offendono le coscienze, che hanno visto questi ragazzi perdere la vita, evidentemente segna la necessità di marcare un punto di svolta. Concludo con un'ultima considerazione. Bisogna far sentire alle famiglie di questi caduti sul lavoro non soltanto l'affetto della comunità nazionale e non soltanto la solidarietà di quest'Aula. Dobbiamo far sentire a queste famiglie che lo Stato esiste non solo quando è vicino alle famiglie, ma quando ha la forza e il coraggio di andare fino in fondo, anche lanciando, dove necessario, qualche monito. La Thyssen

è un segno di arroganza che francamente necessita - lo dico anche al presidente Marini - di essere stigmatizzato, nei modi garbati e nel rispetto di tutti, perché rappresenta una vera e propria provocazione, almeno dal punto di vista di Alleanza Nazionale.

per le vittime di questo incredibile infortunio sul lavoro e anche l'augurio per coloro che stanno combattendo, in condizioni veramente difficili, contro la morte. la morte. Mi unisco a tutti coloro che hanno auspicato un rapido accertamento delle responsabilità, sia nel caso della Thyssen come in quello delle Ferrovie dello Stato, azienda nella quale si è registrato analogamente un infortunio mortale, sia nelle altre aziende in cui purtroppo analoghi infortuni si sono verificati. Devo esprimere subito un sincero apprezzamento per il Ministro del lavoro, perché non si è unito al coro di coloro che hanno voluto leggere strumentalmente, in modo esasperato, questo gravissimo infortunio sollecitando una legislazione emergenziale. Lei, signor Ministro, ha proposto e ottenuto dal Consiglio dei ministri di proseguire nel suo percorso rifiutando una non giustificata legislazione emergenziale per questo l'apprezzo, al di là del giudizio che poi potremo dare sui decreti delegati relativi alla legge delega da poco approvata dal Parlamento. Così come apprezzo che lei abbia subito voluto sottolineare il contesto nel quale questo infortunio si è verificato: non quello di un Paese in cui l'andamento delle statistiche sta peggiorando, ma, al contrario, quello di un Paese che ha registrato, nel corso dei decenni, significative evoluzioni positive da questo punto di vista. Basti pensare ai 4.644 morti nel lavoro del 1963 confrontati con i 1.302 del 2006: sempre tanti, troppi, ma guai a non leggere una tendenza fortunatamente positiva di un Paese che si evolve. Così pure, mi consenta - poiché ho avuto la responsabilità, nel suo Ministero, delle politiche della sicurezza nel lavoro - di ricordare che tra il 2002 e il 2006 gli infortuni sono diminuiti del 6,5 per cento, ma soprattutto quelli mortali sono diminuiti del 12,1 per cento, pari a 176 morti in meno.

Questo è accaduto anche perché, nel corso di questi anni, abbiamo accelerato le politiche per la sicurezza. La stessa legge Biagi contiene numerose tutele prevenzionistiche, che sono state estese a tutti i nuovi lavori, in modo particolare alle collaborazioni a progetto, alle quali si applica il oppure alla somministrazione di manodopera che ha riprodotto la disciplina della legge Treu rafforzandola, o ancora al lavoro intermittente. Ancora, vorrei ricordare che nella stessa legge Biagi si rinviene l'istituzione del documento di regolarità contributiva che è stato richiesto per tutte le opere private e pubbliche in edilizia e che lei ha recentemente voluto estendere ad altri settori; come lì ritroviamo la razionalizzazione dei nostri servizi ispettivi centrali, che abbiamo ricondotto a direzione unitaria e rafforzato con i concorsi per 875 unità che si vanno assumendo, per un totale che dovrebbe portare tutti i servizi centrali del Ministero del lavoro a ben 2.369, quindi ben più del doppio di quanti erano solo fino a poco tempo fa e il totale dei servizi centrali del sistema del Ministero del lavoro a ben 6.403. di una attività che lei ha potuto svolgere - mi consentirà - grazie proprio alla decisione di realizzare quei concorsi e al loro positivo espletamento.

quello cioè di un possibile conflitto di competenze tra amministrazione centrale ed amministrazioni regionali, data l'incerta definizione del Titolo V della Carta costituzionale, che voi avete voluto e che penso non si debba insieme interpretare nel senso di un'esclusiva competenza regionale, tale da produrre una legislazione ancor più difficile da attuare perché diversa da Regione a Regione. Su questo solco lei, Ministro, ha potuto sviluppare un'ulteriore attività, a partire dalla volontà di redigere un Testo unico per il quale le chiedo di accelerare l'adozione di rispetto ai quali avevamo chiesto un tempo più breve di sei mesi, mentre voi avete insistito per nove; la prego, acceleri quest'opera così necessaria, che noi valuteremo

della necessità di sanzioni quanto più proporzionate all'entità delle violazioni, in modo che siano effettive ed utilmente deterrenti. la necessità di un sistema di monitoraggio che ci dica in ogni momento se e per quali patologie o per quali ambienti lavorativi ci stiamo muovendo nella giusta direzione, affinché ciò serva da orientamento

dalla costruzione di un contesto effettivamente ed efficacemente tale da prevenire il verificarsi di lesioni all'incolumità della persona.

della collaborazione tra parti sociali che si realizza attraverso enti bilaterali e organismi con i quali utilmente le parti cooperano in funzione non già del mero rispetto di adempimenti formali, ma del perseguimento di obiettivi sostanziali,

soprattutto nelle piccole imprese (l'esperienza dell'INAIL a questo riguardo è positiva e va resa strutturale). Infine, occorre rafforzare l'esperienza del cosiddetto *bonus malus* nel rapporto assicurativo, tale da premiare i comportamenti virtuosi

invece, ottenere il riconoscimento universale di questo diritto, almeno secondo alcuni criteri essenziali, in modo che la stessa regolazione degli scambi commerciali e la stessa attività dell'Organizzazione mondiale del commercio,

tra i quali anche quello nel quale presto si svolgeranno i giochi olimpici. Per questo la dimensione internazionale è immanente. Noi dobbiamo chiedere di competere con regole sociali si adattano progressivamente allo sviluppo economico, ma che godono nonostante ciò di uno zoccolo fondamentale universalmente riconosciuto nel quale non può non esserci la tutela fondamentale basica della vita del lavoratore. *(Applausi del senatore

signor Ministro, l'esplosione di fuoco che alla ThyssenKrupp di Torino ha investito sette giovani operai, provocando la morte di quattro di loro e il ferimento di altri tre che restano in condizioni disperate, sottolinea tragicamente e drammaticamente le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare quotidianamente tanti, troppi lavoratori nel nostro Paese. Lo scorso anno abbiamo registrato quasi un milione di infortuni, di cui 1.302 mortali. Alla fine di questo anno - i dati in parte già li conosciamo - registreremo sicuramente, purtroppo, un numero di infortuni e di infortuni mortali assolutamente inaccettabile. A tutto questo, inoltre, vanno aggiunte le malattie professionali che nel nostro Paese vengono largamente sottostimate. Con questo quadro e con questa situazione i costi per la mancata prevenzione sono altissimi

Le cause riguardano sovente la mancanza delle più elementari norme di sicurezza. Questo avviene sia nei cantieri edili sia nelle grandi aziende siderurgiche come la ThyssenKrupp e, come abbiamo visto recentemente anche attraverso un'apposita ispezione da parte della Commissione del Senato, l'ILVA di Taranto. Le responsabilità sono delle imprese. A questo riguardo, senza nessuna volontà persecutoria, vorrei ricordare cosa prevede l'articolo 2087 del codice civile.

tutte le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questo dice il codice civile. Certo,

al datore di lavoro l'obbligo di tutelare la salute psicofisica dei propri dipendenti. É stato detto in quest'Aula, anche da parte di chi mi ha preceduto, che ognuno deve fare la sua parte. Sono d'accordo anch'io, tuttavia è necessario che soprattutto ci sia un impegno deciso non formale da parte delle imprese e delle associazioni imprenditoriali ai fini della prevenzione, sollecitando a questo scopo anche la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali. Senza questo impegno

tutte le attività di prevenzione, soprattutto quelle in ambito territoriale e regionale. Queste sono le azioni e gli interventi che devono essere messi in campo se vogliamo effettivamente combattere concretamente la grave piaga sociale che anche oggi giustamente abbiamo

finestra"). Abbiamo così concluso il dibattito sull'informativa urgente del Ministro del lavoro, che ringrazio per la disponibilità, anche nei tempi, dimostrata verso il Senato.

locali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto, il Governo ha approvato il disegno di legge n. 772 per il riordino dei servizi pubblici locali, oggi in discussione, in una delle primissime riunioni del Consiglio dei ministri di questa legislatura e lo ha presentato al Senato il 7 luglio del 2006. Successivamente, il disegno di legge in esame (già presentato come collegato alla manovra per la finanza pubblica per il 2007, poiché rappresenta un intervento suscettibile di determinare un forte e positivo impatto sulla crescita economica e per un nuovo sviluppo dell'Italia),

La discussione in Assemblea è stata tuttavia ripetutamente rinviata a causa della complessità dei lavori di quest'Aula. Ciò ha indotto il Governo, convinto dell'urgenza di introdurre disposizioni indispensabili per frenare il progressivo aumento delle imposte comunali, delle tariffe dei servizi pubblici, nonché della spesa degli enti locali a tutela dei consumatori e dei contribuenti, a presentare un emendamento alla legge finanziaria, diretto a trasformare i contenuti del disegno di legge già licenziato frutto dell'elaborazione avvenuta qui in Senato in Commissione affari costituzionali. Peraltro, proprio oggi l'Aula del Senato è chiamata ad avviare in concreto l'esame del disegno di legge; pertanto, per rispetto delle prerogative del Senato, il Governo ha deciso di non dare corso all'ipotesi di inserire l'emendamento nella legge finanziaria. Tuttavia, nella convinzione dell'assoluta urgenza d'intervenire tempestivamente nella materia, il Governo ritiene opportuno proporre alla valutazione del Senato le stesse disposizioni immediatamente precettive come emendamento al disegno di legge oggi all'esame dell'Aula. Tale iniziativa consentirà, peraltro, al Parlamento di partecipare in maniera diretta alla definizione della riforma. A tal fine, in conformità alle procedure previste per i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, si chiede quindi di rinviare il provvedimento in Commissione referente affinché, in quella sede, possa essere formalizzato l'emendamento annunciato. Il Governo auspica, ovviamente, che il Senato possa pervenire ad una rapida e positiva approvazione della riforma. infine, ringraziare il presidente, senatore Enzo Bianco, il relatore, senatore Giannicola Sinisi e tutti i membri della 1a Commissione per il lavoro intenso, proficuo, approfondito finora svolto che, anche attraverso le numerose audizioni, ha coinvolto gli enti locali e decine di organizzazioni e associazioni sociali ed economiche di categorie del nostro Paese.

attenderemo di conoscere il merito della proposta emendativa che verrà formulata. Con l'occasione, chiedo la cortesia ai colleghi di soprassedere sulle questioni

senza aspettare una delega, così come prevista. Certamente, il problema dei servizi pubblici locali è stato svuotato dall'approvazione, nel decreto fiscale, della norma relativa

Presidente, il Gruppo del Partito Democratico ha molto apprezzato l'intervento del Governo ed il parere reso dal relatore, senatore Sinisi. Ho ascoltato, con molta attenzione, anche gli interventi che si sono succeduti, in particolare quello del collega Eufemi. Signor Presidente, oggi abbiamo letto di una presa di posizione della Presidenza del Senato su cui non possiamo non esprimere, anzi esprimiamo con soddisfazione, un giudizio fortemente positivo. Riteniamo infatti positivo

che aveva una prima previsione di delega, quindi, seppur nell'ambito di princìpi e criteri, si delegava il Governo a fare una norma positiva; poi era corsa voce

con la duplice negatività di aggiungere in finanziaria un carico non proprio e di spogliare il Senato di un lavoro che aveva compiuto. Non possiamo dunque che essere soddisfatti del fatto che il Governo trasformi la delega in norma positiva, perché questo fa guadagnare tempo mette in condizione il Parlamento non di esprimere un parere sul decreto legislativo, ma di approvare la norma positiva, eliminando dubbi e perplessità che pure serpeggiavano nei Gruppi sui contenuti del decreto legislativo

la presa di posizione che ha assunto oggi, a nome di tutti quanti noi e dell'istituzione, il Presidente del Senato, e di questo lo ringraziamo; prendiamo anche atto, con soddisfazione, che il Governo si è, per così dire, ripiegato, e ne siamo contenti,

che, operando in maniera ordinaria, si può anche ottenere un risultato positivo per il Paese e per tutti. Siamo quindi favorevoli a rinviare il in Commissione e nutriamo la speranza che questo possa servire ad un confronto tra i Gruppi che migliori il testo che è stato elaborato, grazie anche all'apporto che darà il Governo con i suoi emendamenti.

dell'ordine del giorno di domani vi è la trattazione del decreto-legge in materia di autorizzazione integrata ambientale, su cui si è registrata una comunanza assoluta di posizioni,

la cui gravità mi sembra inversamente proporzionale all'eco che stanno avendo in Italia. Essa si fonda sul numero delle vittime, sull'individuazione del giorno, sulla rivendicazione, sulla circostanza che sia stato colpito un rappresentante delle Nazioni Unite, come è avvenuto nell'agosto 2003 a Baghdad,

intanto, qual è l'esatta configurazione di questo crimine e poi, visto che è avvenuto sull'altra sponda del Mediterraneo, è importante che il Governo italiano ci aggiorni sulla prevenzione, in chiave di terrorismo islamico ultrafondamentalista, che è arrivato così alle porte dell'Italia.

su un documento del Ministero dell'economia, relativo alla vicenda della privatizzazione di Telecom. Approfitto della presenza del sottosegretario D'Andrea, così sensibile a questi temi, affinché il Ministro dell'economia faccia lo sforzo

un problema così insormontabile; si tratta soltanto di rispettare il Parlamento quando pone problemi di sindacato ispettivo.